Onorevoli colleghi, avverto che l'8a Commissione permanente non ha ancora concluso l'esame in sede redigente del disegno di legge in materia di sicurezza stradale, in attesa del parere della Commissione bilancio. Pertanto, procederemo all'esame dei disegni

*(PD)*. Signora Presidente, prendo la parola perché voglio esprimere, a nome mio personale, ma ritengo anche a nome dei colleghi del Gruppo del Partito Democratico, e probabilmente anche di larga parte dell'Assemblea, fastidio fastidio e amarezza per il livello modesto che stanno assumendo, ormai da vari mesi, i lavori del Senato. Io credo, signora Presidente, che ci si debba ribellare a questo andazzo. Voglio dirle, e l'ho già detto varie volte in quest'Aula, che il nostro calendario è dominato sostanzialmente dalla necessità di convertire decreti-legge: ne aspettiamo tre la prossima settimana e altri due immediatamente dopo. La nostra iniziativa parlamentare è residuale rispetto all'attività di conversione.

e a questo schema di lavoro il Senato si è perfettamente adattato: lo ha assunto come metodo proprio, ordinario di lavoro. di lavoro. Dall'inizio della legislatura, Presidente, noi lavoriamo due giorni alla settimana, e vorrei che la Presidenza del Senato prendesse nota

Le Commissioni, come tutti sappiamo, lavorano negli interstizi dei lavori d'Aula. Lei sa, signora Presidente, e lo sa anche il Presidente Schifani, quante volte il Gruppo del Partito Democratico ha chiesto al Presidente del Senato di Senato di usare la sua influenza sui Presidenti di Commissione per aumentare il tempo di lavoro in quella sede e come

Non dobbiamo meravigliarci se poi sentiamo delle insinuazioni che offendono il Senato, alle quali non voglio dare credito. prego però di riferire al presidente Schifani, che frequenta meno di noi la *buvette*, che urta la sensibilità di chi ha a cuore il Senato sentir dire che questo calendario è stato confezionato per consentire alla Commissione giustizia di lavorare nel tempo in cui l'Aula non lavora, in modo da poter portare avanti l'esame del provvedimento sulle intercettazioni. Io trovo che queste insinuazioni siano insopportabili, perché possono essere pronunciate a causa del modo in cui l'Aula viene governata.

pensavamo che ciò non dovesse accadere e che il provvedimento dovesse tornare in Commissione per poter essere meglio istruito. Così non è stato deciso, ma, a questo punto, il provvedimento deve seguire

dell'Assemblea, presiede tutti gli organi, le Giunte, e da lui dipendono gli uffici. Egli ha tutti gli strumenti per prevedere e prevenire situazioni di stallo dell'Aula; ha tutti gli strumenti per farci lavorare, e questo non accade. Io vorrei pregare lei, signora Vice Presidente, di chiedere al presidente Schifani di usare tutti i suoi poteri per migliorare la qualità del lavoro dell'Assemblea: gli chiedo di non tener conto di pressioni, né dell'opposizione né della maggioranza, ma gli chiedo soprattutto di non far diventare l'Aula del Senato una *dependance* del Governo, come noi stiamo diventando. *(Prolungati Senatore Zanda, la Presidenza non può che prendere atto delle dichiarazioni di carattere generale In merito al provvedimento sulla sicurezza stradale i Capigruppo hanno stabilito un percorso, deferendo il provvedimento alla sede redigente, richiedendo naturalmente un maggiore impegno della Commissione.

Presidente, dopo l'intervento del senatore Zanda, ma su altro argomento, vorrei porre all'attenzione dei colleghi una questione politica che io ritengo di primaria rilevanza e di pieno interesse - immagino - del Senato della Repubblica. Mentre i nostri lavori d'Aula si svolgono con questa calma piatta e queste lunghissime pause, interrotte solo occasionalmente ed episodicamente da qualche rigurgito di attività, quello che accade nelle aule delle Commissioni è sicuramente degno di nota: nelle aule delle nostre Commissioni, sia pure con tempi talvolta molto lunghi e talvolta artatamente accelerati, si discutono questioni importantissime per il futuro del Paese. *(Brusìo).* Vi chiedo scusa, non riesco a parlare. Una di queste è la discussione che si sta tenendo in 7a Commissione sulla riforma dell'università, questione strategica per ogni Paese. Mentre qui, appunto, lunghi soggiorni in Transatlantico e nella *buvette* vengono inframmezzati da rarissimi impegni d'Aula, in Commissione si sta discutendo una riforma dell'università, durante la cui discussione ciascun emendamento che viene presentato dalle opposizioni e che reca un minimo di spesa - dico un minimo di spesa viene regolarmente bocciato perché assistito da un parere della Commissione bilancio, che dice: non c'è un euro. Abbiamo già una severa penalizzazione dell'università operata con le due finanziarie del 2008 e del 2009, una severissima penalizzazione penalizzazione delle risorse. Abbiamo una penalizzazione del Fondo per il funzionamento ordinario dell'università (penalizzazione che pare destinata - ahimè - ad accentuarsi), che oggi impedisce alle università anche soltanto di sapere dove saranno allocate, e per quali fini, le poche risorse rimaste in dotazione al Fondo. In questo modo, come ciascuno di noi sa, essendo ovviamente un referente sul territorio, si è scatenata - ma mi pare anche ovvio - una corsa di tutti i rettori a trovare patronaggi politici per sostenere le proprie università, quindi per un fine pubblico di prima rilevanza ed importanza, così ancora confondendo ciascuno di loro circa quella che sarà la previsione che potranno ragionevolmente fare, perché comunque le università hanno bisogno di redigere un bilancio, di fare un piano per l'anno successivo, di pensare di poter stipulare qualche contratto, addirittura anche soltanto - per quanto riguarda il Fondo ordinario - di poter pagare i dipendenti e di poter organizzare l'acquisto del materiale didattico, oltre che, molto spesso, la locazione di aule nelle quali tenere lezioni. La situazione che si prospetta - lo dicono tutti i colleghi, di maggioranza e di opposizione - è di tale confusione che da qua a due anni non solo le università non virtuose, ma anche quelle virtuose probabilmente chiuderanno. Sono in agitazione i ricercatori, i quali, protestando per la confusione, l'approssimazione e la mancanza di prospettive e di lungimiranza con le quali viene affrontata la loro condizione, non sono oggi disponibili neanche a collaborare all'elaborazione dei piani didattici, che si fondano sulla loro collaborazione per tenere le lezioni, i seminari, le esercitazioni e anche per comporre le commissioni d'esame. In questa situazione due milioni di persone e le loro famiglie non sanno dove sbattere la testa, addirittura non sanno neanche dove indirizzare i sacrifici per l'iscrizione presso quella o quell'altra università, presso quella o quell'altra facoltà. Nessuno sa se privilegiare l'università più vicina, che forse domani chiuderà e che costringerà quella famiglia a rivedere tutti i propri piani finanziari perché il figlio dovrà spostarsi altrove. Non si sa come tutto questo possa assistere (non assisterà in nessun modo) la crescita di una nuova classe dirigente sulla quale noi dovremmo oggi investire: proprio oggi, nella crisi. Mi ha molto colpito, l'altro giorno, una dichiarazione rilasciata dalla *Premier*

in sicurezza, per garantire all'Islanda una classe dirigente in grado di sostenere le difficoltà del Paese nei prossimi 10-20 anni,

del funzionamento dello Stato e - lasciatemelo dire - tra i mille difetti, anche pezzi della sua eccellenza? Questo è il problema. Signora Presidente, le dico con molta chiarezza che il mio Gruppo è talmente esasperato da questa situazione che stiamo considerando il fatto che, di fronte alla nostra richiesta,

ma tante volte sento dire che in questo Paese le leggi sono troppe e che se ne devono abrogare alcune. Il Governo Berlusconi recentemente ha giustamente sottolineato quante norme inutili e superate sono state cancellate. Noi dobbiamo fare buone leggi, utili al Paese:

numerosi provvedimenti riguardanti il lavoro, la scuola, la sicurezza, la lotta alla criminalità, la giustizia, l'economia, con misure apprezzate a tutti i livelli, nazionali e internazionali. L'ultimo l'apprezzamento è di Trichet, che guida la Banca centrale europea, il quale negli interventi fatti nel nostro Paese ha lodato la capacità italiana di affrontare una delicata crisi economica, che la Grecia, la Spagna, il Portogallo e altri Paesi dell'area mediterranea

Più volte - e mi riferisco alle cose che ho sentito poco fa - si è giustamente chiesto da parte di tutti, anche dai colleghi dei Gruppi di minoranza, che le Commissioni abbiano più tempo per svolgere il proprio un apprezzabile e interessante intervento della senatrice Finocchiaro che potrebbe essere svolto tranquillamente nella Commissione istruzione, che si sta lodevolmente occupando, in maniera seria e approfondita, della

da più parti, a dimostrazione del fatto che la pausa non è stata inutile. Poi si può rimanere contrari al testo che ne risulterà, ma se la minoranza ha il diritto di essere contraria, la maggioranza ha il diritto di portare avanti il proprio programma e le proprie leggi in tutti i campi in cui vogliamo esercitare la nostra attività

vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Luigi Palmieri» di Benevento, ai quali diamo il benvenuto.

credo che il tema (che io condivido) sollevato dai colleghi dell'opposizione che mi hanno preceduto non sia legato alla specifica questione dell'andamento dei lavori in Commissione o in Aula questa settimana.

questione che il collega Zanda prima e la collega Finocchiaro poi, oltre agli altri colleghi dell'opposizione, hanno posto, signora Presidente, riguarda il funzionamento del Senato. infatti dirci con assoluta umiltà e con grande franchezza che sono tre mesi che noi facciamo poco o nulla. La maggioranza ha il diritto e il dovere di farsi tutte le leggi che ritiene opportuno fare per garantire il suo programma di Governo, ma questo non significa che quando la maggioranza non ha provvedimenti da presentare si chiude il Parlamento.

che devono essere calendarizzati su proposta dell'opposizione: noi non esaminiamo in quest'Aula nessun disegno di legge di iniziativa di nessuno dei Gruppi parlamentari di opposizione.

è il Ministro che "se la canta e se la suona" in diretta televisiva, a prescindere da ciò che i Gruppi di opposizione dicono. Tutto questo, colleghi, riguarda il funzionamento del Parlamento, che non è solo il luogo in cui esaminare i provvedimenti che afferiscono alla cosiddetta attività d'indirizzo politico: quella è una parte, importante, sempre più importante, ma non esaurisce la democrazia ed il ruolo del Parlamento. Rispetto a questo, il tema che è stato posto è più ampio: non riguarda i tempi di esame, ma la circostanza che, per come sono organizzati i lavori di Commissione, i provvedimenti non hanno il tempo necessario per poter essere esaminati e approfonditi

che questi temi non possano essere liquidati, colleghi della maggioranza, con una sufficienza che rasenta l'irresponsabilità. Questa è la questione sulla quale credo che nel prossimo Consiglio di Presidenza ciascuno, a cominciare dal Presidente del Senato, con chiarezza si dovrà assumere le propria responsabilità.

Gasparri tenda a sminuire l'importanza di quanto segnalato dai colleghi dell'opposizione, noi ci troviamo dinanzi ad un Senato della Repubblica che ormai lavora poco e purtroppo non riesce a incidere sui problemi del Paese. Anche quando le opposizioni fanno esercizio di prudenza e di buona volontà, come sta avvenendo in queste ore per il disegno di legge sulla sicurezza stradale,

io le devo dire che dobbiamo riuscire a far funzionare meglio i nostri lavori nell'interesse degli italiani,

noi siamo perfettamente in sintonia con quanto la presidente Finocchiaro e il presidente D'Alia hanno detto. Chiediamo, e lo facciamo con forza, che il Senato metta in discussione provvedimenti che servano al Paese, ma per definirli. Se non c'è un euro neppure per la sicurezza stradale, come possiamo pensare - lo ricordava la presidente Finocchiaro - di fare una riforma

Signor Presidente, francamente trovo esagerate le critiche dell'opposizione alla nostra maggioranza in riferimento anche alle tempistiche dei lavori d'Aula. Mi permetto di ricordare ai colleghi che la qualità dei provvedimenti non si valuta in base alla velocità d'approvazione in Aula e nelle Commissioni. Il rallentamento dei lavori d'Aula di queste settimane è dovuto al fatto che

sono stati sollecitati, da parte del presidente Schifani e degli Uffici, affinché potessero convocarsi per affrontare i tanti provvedimenti che in questo momento stanno

I provvedimenti che noi affrontiamo in quest'Aula sono gli stessi che affronta la Camera. Anzi, in molti casi il Governo pone la questione di fiducia alla Camera e non al Senato: questo è risaputo.

*Allegato A* DISEGNO DI LEGGE Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003

alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, che prevede la creazione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, concluso a Bruxelles l'8 maggio 2003. Esso consente alle autorità di uno Stato membro che svolgono indagini che svolgono indagini su persone o imprese di conoscere se autorità di altri Stati membri hanno svolto o stanno svolgendo indagini sugli stessi soggetti, attraverso un'informazione sull'esistenza sull'esistenza di fascicoli di indagine. Attualmente, in ambito comunitario, lo strumento-chiave per attuare la cooperazione doganale in ambito comunitario è rappresentato dal regolamento del Consiglio del 13 marzo 1997, che prevede la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola. Tale regolamento prevede l'assistenza e la cooperazione nell'individuazione e nella ricerca delle infrazioni alle disposizioni doganali comunitarie.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo

dati ed il caso in cui la registrazione possa portare pregiudizio all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali.

e tende al potenziamento della collaborazione nelle attività di prevenzione e lotta contro il crimine, estendendo a tutta la materia penale la reciproca assistenza giudiziaria, già in atto per i soli settori della lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga, ai sensi dell'Accordo con il Cile del 1992,

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione: la Commissione, secondo quanto già rilevato con riferimento ad altri provvedimenti di ratifica di accordi internazionali, evidenzia che la modalità di copertura impiegata nel provvedimento non debba essere reiterata per la copertura di futuri accordi internazionali ed invita il Ministero dell'economia e delle finanze ad individuare preventivamente modalità di copertura alternative più conformi alla legge n. 196 del 2009, per le altre ratifiche recanti identica copertura già presentata alle Camere e non ancora discusse».

le questioni attinenti alla lotta al terrorismo. Con il nuovo testo le parti si impegnano ad estendere la loro collaborazione ad una serie di atti giuridicamente impegnativi, che tuttavia non contrastano né con le norme

di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo,

legge n. 2110** Il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, riguarda l'accordo multilaterale tra Unione europea e numerosi Stati limitrofi per la creazione di uno spazio aereo comune.

nel presupposto che agli oneri del provvedimento si provvederà con risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

stiamo parlando della ratifica e dell'esecuzione dell'Accordo multilaterale della Comunità europea ed i suoi Stati membri con tutti i Paesi dei Balcani occidentali. Volevo soltanto far rilevare, visto e considerato che si tratta di tutti Paesi con cui l'Italia intrattiene importanti

ne è stata una prova recente anche il blocco che è intervenuto nei cieli dovuto alla

*(PD)*. Signora Presidente, in data 18 febbraio 2010 (non sembri una coincidenza con i temi che ha trattato autorevolmente la Presidente del nostro Gruppo) insieme alla senatrice Leddi

dati vigenti del Ministero; quindi rifletteva una realtà preesistente e pur tenendo conto dei parametri ministeriali registrava una situazione drammatica,

Chiediamo quindi che doverosamente il Ministero risponda a queste domande che erano precise ed istruite e che aggiungono allo stato delle cose esistenti una crescente esigenza di risposta.

Presidente, mi rivolgo a lei. Il 4 maggio davanti a Montecitorio... *(Brusìo).* PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, non riesco a sentire le richieste dei senatori.

Chiedo, Presidente, come mai non venga riconosciuto a queste persone, precarie da anni, nemmeno il loro impegno nel tutelare le nostre famiglie e i nostri territori. Chiedo quindi al Ministro le ragioni per cui, pur essendovi una grande carenza di organico nei Vigili del fuoco queste persone restano dei precari e inoltre sono costrette a manifestare per aver riconosciuto un giusto diritto. Inoltre, domando al ministro Maroni quali provvedimenti intenda chiedere al riguardo e quali sono i tempi per risolvere questo gravoso problema. I Vigili del fuoco hanno manifestato, e con loro c'era anche il Partito Democratico. Colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto tecnico industriale minerario «Giorgio Asproni» di Iglesias, ai quali diamo il benvenuto.

so che il ministro dell'economia Tremonti sulla crisi dei mercati andrà a riferire alla Camera nei prossimi giorni. Non è la prima volta che noi poniamo all'attenzione del Senato, come Gruppo Italia dei Valori, la questione di una crisi che fa paura all'Europa. Euro e borse sono andati a picco ieri: sulle piazze europee sono stati bruciati 144 miliardi di euro; Milano ha perso il 4,70 per cento; Wall Street il 2,38. Oggi si sono verificati dei tumulti, degli scioperi e ci sono stati tre morti in Grecia. Penso che i Governi democratici debbano porsi questo problema, perché mentre la Grecia e parte dell'Europa bruciano per diretta responsabilità dei banchieri centrali, collusi con politici ed alcuni Capi di Governo, Paesi come la Germania hanno utilizzato i secchi d'acqua non per spegnere l'incendio ma per farsi la doccia ed arrivare puliti ai funerali dell'euro. Noi dobbiamo verificare quello che sta accadendo. La politica ed i Governi hanno delegato troppo all'oligarchia, che mette in atto una potenza di fuoco senza precedenti per condizionare i Governi democratici e per attentare alla sovranità degli Stati. c'è la Spagna (abbiamo visto oggi la fuga dei capitali), il Portogallo e anche noi, benché siamo messi meglio degli altri, abbiamo un debito pubblico che rischia di fare paura (30.000 euro ogni singolo cittadino). Quindi, signora Presidente, ritengo che dovremmo portare all'attenzione dell'opinione pubblica tale questione, perché non si può permettere la dissoluzione della civiltà giuridica e dei Governi democratici, una dissoluzione che è voluta dalle banche di affari, dalle agenzie di *rating* e da questi signori collusi, che per la loro avidità di guadagno seminano miserie e macerie nel mondo globalizzato. Si tratta di una questione che anche il Senato della Repubblica dovrebbe affrontare, e mi auguro che il ministro Tremonti venga anche in quest'Aula,

per questi disastri che ha combinato. Signora Presidente, mi devo associare alla collega Negri per richiamare altre numerose interrogazioni che riguardano scuola e università, ma mi fermo all'università perché le situazioni stanno diventando sempre più drammatiche proprio in costanza di un grande impegno del Senato per la riforma universitaria. Vorrei pensare che il presidente Gasparri è troppo intelligente per non aver capito il senso dell'intervento della mia presidente, che era di grande allarme sul fatto che stiamo facendo una riforma importantissima che non ha alcun finanziamento; anzi - a detta del Ministro dell'istruzione - non sarà chiesto nemmeno un euro in più al Ministro dell'economia per situazioni come quelle appena ricordate dalla collega Negri. Allora, credo che, con il con il desiderio di collaborare, possiamo chiedere ai Ministri di rispondere alle nostre interrogazioni, perché potrebbero essere la sede opportuna per verificare questo fatto semplice: se una riforma così importante non viene finanziata, diventa una presa in giro perfino continuare a discuterne. Credo che la presidente Finocchiaro volesse dire che il nostro Gruppo non vuole partecipare a questo inutile *show* chiedendo una riforma che non si farà. Pertanto, potremmo addirittura pensare di non partecipare ai lavori. È urgente quindi che i Ministri vengano a rispondere in Aula.